nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

confesso la mia emozione: mai nella vita, quando ho cominciato la mia attività politica, avrei pensato di sedere sui banchi del Governo, ma neanche sui banchi del Parlamento. Sento forte l'onore, l'onere e la responsabilità. È il mio primo intervento, quindi ringrazio voi per l'attenzione

ringraziare l'ex procuratore di Venezia, Carlo Nordio, che oggi ha scritto un articolo che mi ha confortato, dal titolo «Diritto e diritti: la lezione che nessuno può dare al nostro Paese», che mi impone di dire che intervengo a nome di un Governo e di una maggioranza, ma che arrivo ad avere l'ambizione di parlare a nome di un popolo che in termini di generosità, volontariato, accoglienza e solidarietà non Il problema non è il *derby* Italia-Francia dei mondiali, che peraltro ci vedono esclusi, ma che la nostra storia

FdI).* Carlo Nordio, come dicevo, scrive: «Il diritto internazionale, come tutto il diritto, non è una scienza esatta», quindi abbiamo letto tutto e il contrario di tutto. Aggiunge che «l'emigrazione, da fenomeno relativamente modesto e controllabile, è diventata un'invasione, gestita da criminali», e conclude ricordando che il nostro nuovo Governo «avrà molti difetti» - vero - ma in questo momento, su questo tema, «si sta comportando con coerenza e dignità», alle quali aggiungo l'umanità.

Non abbiamo avuto risposta: evidentemente, l'emergenza non era così emergenziale. In questo momento, la nave Aquarius, con due navi della Marina e della Guardia costiera, sta navigando serenamente verso le acque di un Paese che si è detto disponibile

i respingimenti alla frontiera tra Italia e Francia hanno visto rispedire a casa nostra 10.249 esseri umani, compresi donne, bambini e disabili. Sulla base degli accordi sui ricollocamenti del 2015, la Francia si era impegnata ad accogliere 9.816 immigrati in tre anni, invece di 9.816 immigrati, ne ha accolti 640. Quindi, chiedo al presidente Macron di passare dalle parole ai fatti e di accogliere domani mattina i 9.000 immigrati che si erano impegnati ad accogliere *(Applausi dai generosità concreta, non solo a parole. Ricordo che l'Italia, in questo momento, è il secondo Paese per accoglienza in tutta Europa: quindi, di questo stiamo parlando. Stiamo verificando i costi e i tempi, perché il problema su cui dovremo lavorare sono i costi e i tempi: chi mi ha preceduto ha fatto un buon lavoro e noi non siamo qua per smontare il buon lavoro fatto da altri, ma cerchiamo semplicemente di fare un lavoro ancora migliore. Non siamo particolarmente intelligenti, ma prendiamo atto di quanto è stato fatto di positivo e vedremo di fare ancora meglio. Quel che non funziona e su cui, evidentemente, chi mi ha preceduto non è stato abbastanza fortunato ed efficace, sono i tempi di identificazione, perché dal momento dello sbarco alla chiusura del percorso, compresi i ricorsi, passano fino a circa tre anni, che è un lasso di tempo inaccettabile e incomprensibile. Per quanto riguarda i costi per ogni singolo richiedente asilo, ricordo che i francesi spendono 25 euro al giorno, a cui aggiungono in qualche caso quattro euro di *pocket money*, i tedeschi 26 euro, i croati 25 euro, gli austriaci 23 e via dicendo. Quindi, cercheremo di portare i costi di questa immigrazione, per noi difficilmente sostenibili, al livello dei Paesi nostri simili in Europa. Non si vede perché dobbiamo spendere 35 euro per garantire servizi che in altri Paesi comportano una spesa molto minore. settimana prossima avrò l'onore di incontrare 250 ragazze e ragazzi formati per far parte delle nuove commissioni di identificazione e riconoscimento, per accelerare ancor di più i tempi di di distinzione tra i rifugiati e coloro che rifugiati non sono. Ricordo i numeri - che amo - di questo 2018: fra le 42.000 domande esaminate c'è un rifugiato politico - è stato riconosciuto come tale - in sette casi su 100. Se aggiungiamo i quattro casi su 100 di protezione sussidiaria, arriviamo a un 11 per cento. C'è una maggioranza assoluta delle domande che viene respinta, perché priva di qualsiasi fondamento. Il problema è che dietro c'è un *business* e lo diciamo ad alta voce: il 99 per cento delle domande respinte è oggetto di ricorso e c'è il *business* degli avvocati d'ufficio, che fanno milioni di euro sulla pelle di questi disgraziati e occupano le aule dei tribunali. Quindi, anche su questo occorre fare qualcosa. Arrivo alla relazione che i miei uffici mi avevano preparato.

Il giorno 9 giugno 2018 si sono verificati, all'interno dell'area di responsabilità dichiarata della Libia, sei eventi distinti per i quali il centro di coordinamento delle capitanerie di porto con sede a Roma ha ricevuto le prime richieste di soccorso. A seguito di tali richieste, il centro di coordinamento di Roma ha provveduto a interessare l'autorità libica. Il primo problema è che, sebbene la Libia abbia ratificato la Convenzione di Amburgo del 1979 e abbia recentemente dichiarato la propria area di ricerca e salvataggio, non ha assunto il coordinamento dei sei Va peraltro precisato che, con il sostegno delle capitanerie di porto italiane, la Libia sta gradualmente procedendo ad attivare un proprio centro di coordinamento soccorsi. Stiamo lavorando perché io personalmente, entro il mese di giugno, possa andare in Libia per cercare di garantire eguaglianza di diritti e di doveri su entrambe le sponde del Mediterraneo. Dopo il "no" libico è stata altresì contattata l'autorità Search and Rescue (SAR) maltese, in quanto centro di coordinamento e di soccorso responsabile per l'area immediatamente limitrofa a quella degli eventi; tuttavia neppure la predetta autorità maltese ha assunto la responsabilità del coordinamento, come sono abituati a fare da anni. Il fatto che il Governo abbia alzato, per una volta, la voce probabilmente metterà i maltesi di fronte alle loro responsabilità al fine di aiutarci a salvare vite umane. umane. Il centro di coordinamento di Roma ha quindi dovuto proseguire nella direzione delle operazioni di soccorso per i sei eventi sopramenzionati. L'attività di coordinamento delle operazioni ha portato al salvataggio di 629 persone che sono state riunite sulla nave Aquarius. Aquarius. Completate le operazioni di salvataggio, la nave Aquarius cominciava la sua navigazione verso Nord e, una volta raggiunta l'area SAR maltese, al fine di garantire il prima possibile assistenza ai migranti,

Sul punto è opportuno specificare che la nave Aquarius, alle ore 12 di domenica 10 giugno, quando si trovava a circa 64 miglia nautiche a Sud dell'isola di Malta, ha manifestato problemi di sicurezza a bordo e quindi ha chiesto alle autorità maltesi di poter sbarcare sull'isola le persone soccorse. In attesa di tale riscontro più volte sollecitato e che perdurava per l'intera giornata di domenica 10 giugno, la nave Aquarius continuava a permanere nelle aree di competenza maltese. Nelle prime ore della notte dell'11 giugno, il comandante della nave comunicava al centro di coordinamento di Roma il peggioramento della situazione sanitaria, nonché lo scarseggiare di risorse alimentari. Ancora sollecitati nella mattinata dell'11 giugno, con una comunicazione ufficiale al centro di coordinamento di Roma, Malta negava la propria competenza sull'evento in questione: se ne fregava. In attesa In attesa di determinazioni in merito all'individuazione di un porto sicuro di sbarco (POS), la nave Aquarius, che stazionava nella zona di ricerca e soccorso maltese, è stata costantemente affiancata da motovedette della Guardia costiera italiana, con personale medico imbarcato per fornire eventuale assistenza sanitaria. È stata altresì rifornita delle derrate alimentari e di quant'altro necessario per tutte le persone a bordo. Sottolineo, come ho già detto, che è stata offerta al comandante della nave Aquarius per ben due volte, alle ore 12,11 e alle ore 14 dell'11 giugno, la disponibilità delle autorità italiane, su mia indicazione, a far sbarcare sul territorio nazionale le persone eventualmente bisognevoli di assistenza sanitaria, quali ad esempio le donne incinte e i bambini; disponibilità che non è stata accolta dal comandante dell'unità. nota la differenza tra la realtà virtuale e la realtà reale, tra quello che si leggeva sui siti Internet, sui giornali e sui *social*

Nelle prime ore del pomeriggio dell'11 giugno il Governo spagnolo comunicava la propria disponibilità allo sbarco dei 629 migranti presso il porto di Valencia; disponibilità formalizzata successivamente, alle ore 22,48 dello stesso giorno. Io ringrazio gli amici spagnoli,

16.000 contro 170.000. Ringrazio il buon cuore del presidente Sánchez, il quale ha ampio margine per esercitare la sua generosità e la sua accoglienza anche nelle settimane a venire*,* visti i numeri da cui partiamo*. Il comandante rappresentava che, per effettuare il viaggio in sicurezza, la nave Aquarius non avrebbe potuto ospitare a bordo più di cento

per assistere l'Aquarius e prendere a bordo 250 persone sull'Orione e 273 sulla Dattilo e accompagnare per un viaggio tranquillo e sicuro verso il porto di Valencia la suddetta nave Aquarius.

nell'anno scorso, grazie a operazioni utili e intelligenti di chi mi ha preceduto, sul fronte della riduzione del numero degli sbarchi, cosa alla quale cercherò di lavorare ancora di più. Ci sono alcune stranezze: la prima etnia per sbarchi quest'anno è rappresentata da circa 3.000 cittadini tunisini. Mi premurerò di incontrare il prima possibile anche il mio collega tunisino, perché mi sembra che la Tunisia risulti un Paese libero, dotato di autonome istituzioni, non è vittima di guerre, pestilenze o carestie, quindi cercherò di portare tutto il conforto e l'aiuto necessario da parte del popolo italiano al popolo tunisino per far sì che questi ragazzi e queste ragazze possano crescere e cercare un lavoro e una vita nel loro Paese, piuttosto che mettersi su un barcone. tre, quattro o cinque pagine, ma preferisco dedicare il tempo a voi, piuttosto che a leggere numeri. Ci tengo a dire che in queste ore ho sentito tanti colleghi europei. Leggevo che l'Italia è isolata. Penso che non siamo mai stati così centrali e così ascoltati come in queste ore. Ho parlato con il collega tedesco, con il quale abbiamo condiviso che occorre tornare a ragionare di protezione delle frontiere esterne italiane come frontiere europee e non solo italiane. Non possiamo essere gli unici a fare quello che meritoriamente facciamo nel Mediterraneo, sopportandone costi economici e costi sociali. Se l'Europa c'è, batta un colpo adesso o taccia per sempre. Noi gliene abbiamo dato l'occasione e l'opportunità. Ho sentito il collega francese, quello ungherese, incontrerò il collega austriaco, ho sentito ambasciate di diversi Paesi, dalla Tunisia alla Libia. Quindi c'è un'attenzione che non c'è mai stata; sta a noi adesso giocarci le carte in maniera propositiva, non solo negativa. Il regolamento di Dublino oggi evidentemente va superato. Hanno provato a imporci una norma che avrebbe ulteriormente aggravato la situazione in Italia, con una permanenza fino a dieci anni di ulteriori migranti, senza alcuna possibilità di essere accolti accolti in altri Paesi. Abbiamo concordato un no costruttivo e penso che con il collega tedesco e con il collega austriaco - visto che dal 1° luglio la competenza e la presidenza europea sarà dei colleghi austriaci - proporremo una nostra iniziativa, sul fronte interno e sul fronte esterno. ho avuto un peso notevole sulle spalle. La critica politica ci sta, è giusta, è sana. Il mio obiettivo è salvare vite; il mio obiettivo è far sì che questi bimbi possano crescere nella migliore maniera possibile, senza scappare dai loro villaggi e dalle loro città per mettersi su gommoni, che ormai i delinquenti del *business* del traffico di esseri umani fanno partire già sgonfi, perché tanto c'è qualcuno che va a recuperare questi disgraziati. Vedremo nelle prossime ore. Stanno sbarcando migranti raccolti dalle navi delle autorità militari italiane. È tempo che gli Stati tornino a essere Stati. Non è possibile che siano associazioni private finanziate da chissà chi a imporre tempi e modi dell'immigrazione. Basta guardare, infatti, da dove arrivano alcuni finanziamenti, anche se questo tema sarà oggetto di una prossima informativa. Io adoro ogni tipo di generosità e di volontariato, sono donatore di sangue e di organi, ma quando leggo che dietro a qualche organismo c'è la Open Society Foundations di George Soros, qualche dubbio inizia a venirmi

Chiudo con una riflessione: «Ama il prossimo tuo come te stesso». Giusto. Il mio prossimo, quindi, sono donne e bambini che fuggono della guerra e che sono le prime vittime della confusione che stiamo vivendo. Quei pochi ragazzi, donne e bambini che scappano dalla guerra devono avere in casa nostra casa loro e non possono essere mischiati ad una immigrazione clandestina che porta semplicemente allo scontro sociale. Però «ama il prossimo tuo come te stesso» significa anche amare i milioni di italiani che in silenzio hanno perso casa, lavoro e speranza. che hanno perso casa, lavoro e speranza. Quindi, con tutti i miei limiti e tutti i miei difetti, farò tutto quello che è umanamente possibile per dare voce ai rifugiati veri, agli immigrati regolari e per bene che vengono qui per costruire per se stessi e per i loro figli un futuro, rispettando la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni, e soprattutto farò di tutto perché a questi italiani che hanno perso la speranza, questa possa tornare e a ciò dedicherò tutti i miei prossimi anni da Ministro ma soprattutto di vita, onorato di poterlo fare a disposizione del popolo italiano. Grazie a tutti.

932 persone che si aggiungo alle tante che abbiamo salvato in tutti questi anni. Apro una parentesi e la chiudo, solo per una piccola correzione al Ministro che ha dimenticato di dire che diverse delle persone che erano sulla nave Aquarius sono state ivi trasportate da imbarcazioni della Guardia costiera italiana.

932 persone che sono sbarcate sono l'ultimo tassello di una catena. Vorrei dire alle autorità estere, agli Stati amici, all'Europa: i Governi passano, gli Stati rimangono. Noi non possiamo non privilegiare sempre, e lo dico anche a voi in quest'Aula, uno spirito di continuità istituzionale, perché su questo principio è fondata la Repubblica. L'Italia non può accettare lezioni e gli insulti che i francesi ci hanno rivolto in queste ore,

signor Ministro, lei deve sapere che nessuna polemica politica, anche aspra, che ci potrà dividere nei prossimi anni, ci potrà portare ad assumere un connotato e una veste anti-istituzionale e anti-italiana. Mai, perché questo contrasterebbe con la nostra storia. Tra l'altro, è inutile che si ricordino i comportamenti inumani che i nostri colleghi hanno avuto a Bardonecchia o a Ventimiglia, ma io vorrei aggiungere un aspetto importante: in questi mesi, c'è stato un traffichìo che non mi è piaciuto, in Libia, da parte delle autorità francesi, autorità francesi, che sono le stesse che negli anni scorsi hanno lavorato, probabilmente sottobanco, per una tripartizione della Libia, mentre i Governi Renzi e Gentiloni Silveri lavoravano per garantire l'unità della Libia e aiutare il Governo legittimamente insediato dalle Nazioni Unite. si tratta solo dell'inumanità di certi respingimenti, ma anche di un lavoro sottobanco che noi dobbiamo portare all'attenzione della comunità internazionale e dell'Europa, perché non è possibile che i principali attori o *player* europei giochino parti diverse nella stessa commedia su uno scenario come quello libico. Non è un caso

Noi siamo stati lasciati soli, lo ha ricordato la signora Merkel. Signor Ministro, lei fa benissimo a parlare con tutti, siamo stati lasciati soli da tutti. Lei ha ricordato i dati della Spagna, io vorrei ricordare gli atteggiamenti delle autorità di Visegrád, quando, davanti all'idea della redistribuzione sono stati i primi a dire: «In casa nostra no». *(Applausi dal Gruppo PD).* Ora, noi oggi cerchiamo alleanze con costoro, è vero che San Paolo si è convertito sulla via di Damasco, io mi auguro che lei sia più bravo di chi ha convertito San Paolo, ma

secondo punto: la continuità istituzionale. Le posso dare un suggerimento? Io sono un vecchio, qualcuno dice anche troppo, ma tollerate anche gli anziani perché la società è fatta di giovani e anziani (dicevano che si difendono le città con le armi dei giovani e con i consigli degli anziani). Le consiglio di offrire un caffè al suo predecessore, proprio nello spirito di continuità istituzionale a cui ho fatto riferimento, perché perché c'è un portato di esperienza di chi, a mio parere, ha operato bene - perché le statistiche dimostrano che il suo predecessore ha operato bene - che non può essere disperso oggi.

ma smettiamola di fare la campagna elettorale, tutti insieme, sulla pelle di questi disgraziati, perché questo non porterà alcun vantaggio all'Italia, al Governo che lei autorevolmente rappresenta, ma anche all'opposizione. Questo è un tema troppo importante per fare su di esso una campagna elettorale permanente.

Al primo posto in questa scala di valori - non dimentichiamocelo mai - viene sempre il principio dell'umanità che si sostanzia nel rispetto della vita, delle persone e della dignità umana.

nel momento in cui ha chiesto il soccorso. Questo avremo possibilità di vederlo dopo. Su questi punti - lo sa meglio di me - e su questa vicenda

Ciò significa che non siamo consapevoli delle responsabilità dell'Europa? Altroché, se ne siamo consapevoli. Abbiamo assistito in tutti questi anni a un rimpallo di responsabilità e

accettare la decisione che lei ha assunto. Chiedere che l'Europa inverta la rotta, modifichi le regole sbagliate, riveda il Trattato

come Paese. Per il cinismo che è stato dimostrato in questa occasione - torno a ripeterlo, il cinismo - oggi rischiamo di non mettere il nostro Paese nelle condizioni di costruire le migliori alleanze per una vera riforma delle regole europee.

d'accordo sulla ricostruzione fatta dal Ministro dell'interno, quindi non mi dilungherò perché l'applauso che gli abbiamo riservato, da forza di opposizione, dimostra che quando il Governo si comporta in maniera corretta troverà sempre il sostegno anche di chi non sostiene questo Esecutivo. Ed ho visto con piacere che la stessa accoglienza è stata manifestata da tutto il centrodestra, anche da Forza Italia, oltre che da coloro che sono al

veramente verificato - lo dico in assoluta buona fede - se a un aumento delle partenze corrisponda un atto umanitario o se invece, tirando le somme di quello che è avvenuto in questi anni, ci si sia resi conto che, al di là delle buone intenzioni (che io non voglio escludere in partenza) a tale aumento sia corrisposto un aumento dei morti.

tutta d'oro, tutta d'argento. Signor Presidente del Senato, signor Ministro, senatori, cosa chiede Fratelli d'Italia? Pensa che questa ottima scelta del Ministro possa essere la soluzione? No, questo è un segnale importante all'Europa, agli altri Paesi; non può essere la soluzione.

in Italia. Signor Presidente, riteniamo che allora la soluzione (e se c'è bisogno di fare leggi, facciamole), che peraltro è di minore rischio per chi drammaticamente viene raccolto da quelle navi, sia fare entrare le navi nei porti in futuro,

E magari denunciare per tratta di uomini, donne e bambini coloro che si prestano a trasportarli, magari in accordo con gli scafisti. Lo dice La Russa? Colleghi, l'allarme non l'ha lanciato Salvini non l'ha lanciato Salvini né La Russa, Fratelli d'Italia o la Lega. L'allarme l'ha lanciato una delle persone più stimate nell'ambito della magistratura, di cui ho l'onore di conoscere il percorso: il procuratore capo di Catania,

Fratelli d'Italia si aspetta che il percorso prosegua nel rispetto delle vite umane e nel desidero di aiutare chi possiamo aiutare, ma nella fermezza che ciò servirà ad aiutare chi ne ha bisogno e a rendere più tranquilli i cittadini italiani che ne hanno diritto.

ciò non ci esime dal dare un giudizio politico. Ministro Salvini, la vicenda della nave Aquarius sintetizza bene uno stile di Governo mirato più a continuare i toni roboanti della campagna elettorale, che a risolvere davvero i problemi degli italiani, come lei dice di voler fare. Problemi che quanto più sono complessi (la vicenda delle emigrazioni, dopo un periodo di tensioni, turbolenze e guerre che hanno riguardato il Nord Africa e il Medio Oriente, rientra nel novero dei problemi molto complessi), problemi molto complessi), tanto più necessitano di strategia e non di azioni e proclami propagandistici. Con la cosiddetta chiusura dei porti alla nave Aquarius, lei si è voluto presentare come l'uomo forte, ma in realtà ha manifestato una grande debolezza. Il muro da lei eretto contro più di 600 persone in grave difficoltà non ha fermato gli sbarchi. Il tema non è quello di fare azioni eclatanti, bensì come si continua a governare i flussi. Lei lo sa bene, perché i dati non sono manipolabili, neanche dalla propaganda. Con l'azione del ministro Minniti i flussi degli arrivi sono diminuiti dell'80 per cento, in generale, e dell'85 per cento per quanto riguarda quelli provenienti dalla Libia. Perché, allora, la chiusura dei porti? I porti si chiudono solo in casi eccezionali, di vera grande emergenza per il Paese. Lo scorso 10 giugno, a urne aperte, quando lei, ministro Salvini, ha ingaggiato la battaglia con Malta, non c'era alcuna emergenza migranti. I numeri degli arrivi erano già stati assai contenuti da chi l'ha preceduta. Perché lo ha fatto, allora? Prima ha parlato di *business*, si è espresso con parole offensive nei confronti della Tunisia, dicendo che la pacchia è finita, e poi ha chiuso i porti. Il suo gesto è stato solo simbolico e propagandistico; una crudeltà inutile, simbolica e inumana.

E non dica che lo ha fatto perché l'Unione europea si rendesse conto. Che cosa sarebbe successo se la Spagna non avesse dato disponibilità all'accoglienza? La disponibilità data dal Governo spagnolo non è un suo successo. Il Governo Sánchez ha dato dimostrazioni di solidarietà non alle sue posizioni, ma alle persone stipate su quella nave, lasciate sole in mezzo al Mediterraneo. Il muro da lei eretto non ha fermato gli sbarchi (ne è prova ciò che sta avvenendo stamattina a Catania), ma ha isolato l'Italia. Le sue parole e le sue azioni stanno isolando l'Italia in Europa e nel mondo; isolandola perché dalle nostre azioni prendono le distanze la Spagna, la Francia, la Tunisia. Vedremo come procederà la collaborazione che con la Libia avevamo attivato e che aveva dato frutti importanti. Ha ricevuto sostegno solo da alcuni *leader* del gruppo di Visegrád, peraltro quegli stessi *leader* che si rifiutano di accettare i ricollocamenti europei. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Neppure un rifugiato avente diritto è stato accettato da chi ora plaude alla sua azione. Senza una politica per l'Africa, senza i rimpatri, senza i ricollocamenti, cosa rimane di una strategia politica di governo dei flussi, che era un patrimonio dell'Italia, non di un Governo, non di una maggioranza, ma dell'Italia, proprio quella di cui lei ha parlato? *(Commenti dai Gruppi ma è una direzione senza strategia, è un'azione inconcludente; ma è un'azione rivelatrice. Noi avevamo chiesto questa mattina al *premier* Conte di essere qui in Aula. Un Presidente del Consiglio che fino ad ora non ha speso una parola sulla questione di attualità più scottante per il nostro Paese e che avrebbe dovuto fare sintesi dell'azione dei Ministri. La chiusura dei porti, come lei ben sa, non spetta a lei, ma spetta al ministro delle infrastrutture Toninelli. Nulla dal *premier* Conte, silenzio assordante. Ne dobbiamo dedurre che è il Governo Salvini e non Conte quello che oggi guida l'Italia. Ha questa grande responsabilità? Bene, allora mi dica: è vero, l'Europa deve e può fare di più, ma per ottenerlo si possono usare degli ostaggi? Perché questo è quello che lei ha fatto: lei non ha esitato a prendere in ostaggio più di 600 persone inermi e disperate, per farsi sentire al tavolo europeo.

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, il caso Aquarius segna senza dubbio un cambio di rotta della politica italiana sulla gestione dei flussi migratori. L'attuale Governo ha dato al Paese intero un segnale chiaro di cambiamento. E questo è il primo passo del Governo del cambiamento. Quante volte abbiamo assistito, in questi anni, a vertici europei che parlavano di leale collaborazione, di solidarietà (per la gestione dell'immigrazione soprattutto), di una politica comune? Quante strette di mano, quante parole al vento, per fingere l'esistenza di un'Europa unita e solidale! I cittadini italiani alle scorse elezioni hanno capito di essere stati presi in giro da Governi che si sono dimostrati incapaci di passare dalle parole ai fatti nei rapporti con l'Unione europea, in particolare sul tema dell'immigrazione. L'Italia L'Italia è stata abbandonata ai suoi doveri; la frontiera europea ormai si è spostata a nord dell'Europa. Qualcuno ha definito vomitevole l'azione politica di questo Governo e questo qualcuno, la Francia, è proprio quel Paese che ha chiuso le frontiere di Ventimiglia e che è responsabile del vergognoso fatto di Bardonecchia, quando le autorità francesi hanno chiuso le porte a una donna nigeriana incinta e malata, poi morta dopo il parto. Proprio quel Paese Proprio quel Paese si è affrettato a smentire la disponibilità ad accogliere la nave Aquarius la scorsa mattina. Noi non Noi non accettiamo lezioni di civiltà dalla Francia o da qualunque altro Paese, neanche dalla Spagna delle barriere di Ceuta e Melilla, e non accettiamo lezioni di umanità da forze politiche bocciate alle urne dagli elettori e che hanno ridotto questa Nazione allo stato attuale, specialmente in tema immigrazione. La gestione incontrollata dei flussi migratori ha portato, negli ultimi quattro anni, a oltre 15.000 morti in mare e ci è costata miliardi e miliardi di euro: quanto accaduto non ha assolutamente nulla a che vedere con l'immigrazione che ho vissuto io. Bisogna essere chiari: l'unico modo per non far morire in mare queste persone è non farli partire attraverso quei tunnel della morte.

La criminalità organizzata nel Nord Africa continua a gestire la tratta degli esseri umani e noi non possiamo continuare né a gestire da soli questo fenomeno,

Questo Governo, a differenza dei Governi precedenti, chiama l'Europa ai suoi doveri, svegliando la coscienza della comunità internazionale e chiedendo con i fatti e a gran voce che l'Italia non sia lasciata da sola ancora una volta: chissà perché, quando c'è qualcuno che chiede o decide di cambiare davvero le cose, tutti criticano senza avanzare mezza soluzione al problema. FdI)*. Ministro Salvini, apprezziamo profondamente il suo equilibro, la sua saggezza, il suo coraggio e il buonsenso, con i quali ha iniziato finalmente a risolvere questo problema.

finalmente l'Italia ha un Governo che ha a cuore la sicurezza e il benessere del suo Popolo nel rispetto della dignità umana. Io non voglio essere complice del nuovo schiavismo moderno. *(Applausi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro dell'interno, il Gruppo di Forza Italia condivide, dalla prima all'ultima, le parole che lei ha pronunciato in quest'Aula e non abbiamo difficoltà a ribadire che noi che non abbiamo votato la fiducia a questo Governo, al quale molte cose avremmo da criticare (ma lo faremo quando ci arriveremo), siamo legati al programma che anche lei con noi ha sottoscritto sull'immigrazione: i punti che il centrodestra ha proposto agli italiani. Li ricordo a noi stessi in sintesi: la ripresa del controllo dei confini; il blocco degli sbarchi e i respingimenti assistiti; un piano Marshall per l'Africa; il rimpatrio dei clandestini e l'abolizione di quel singolare istituto della protezione umanitaria, perché i profughi sono profughi e i clandestini sono clandestini e questa terza via italiana non va Noi siamo vincolati a quel programma: se il Governo agirà su quello che è un programma che anche lei, Ministro, conosce e ha sottoscritto, la nostra posizione sarà chiara e trasparente, senza dover essere ipocriti.

Se gli sbarchi sono diminuiti, e non abbiamo difficoltà a riconoscere la *Realpolitik* che anche Minniti ha praticato, resta tuttavia l'azione di partito di cultura di governo che Forza Italia ritiene di realizzare in ogni fase della vita politica italiana

Grazie a tutti. le navi italiane che stanno in zone in cui il soccorso deve essere fatto dai maltesi, dai libici e da altri, rischiano di riempirsi di clandestini e di sbarcare a Catania, come sta avvenendo in questo momento con una nave della Guardia costiera. Quelle navi, se non servono a combattere il traffico, le mandi a Livorno, a Venezia, a Ventimiglia

hanno detto altri colleghi, ma lo voglio ribadire. Non le accettiamo dalla Spagna, che sparava a Gibilterra; non le accettiamo dalla Francia, che da Ventimiglia a Bardonecchia ha agito come sappiamo. Noi non vogliamo le crisi emetiche della Francia; vogliamo le frontiere ermetiche dell'Europa.

Noi prendiamo lezioni dai Governi di centrodestra guidati da Berlusconi, che hanno attuato la *Realpolitik* sul fronte dell'immigrazione: lei, Ministro, ha tre o quattro Gheddafi con cui deve parlare: i sindaci del Maghreb, Sarraj, Haftar. Non sarà facile la sua missione in Libia, ma dovrà farla. E allora, noi prendiamo lezioni da quei Governi e da quelle politiche che rivendichiamo e lei e il suo partito le avete condivise con quei Governi e quindi come noi può esserne orgoglioso.

a portare solidarietà. Quindi, a proposito di porti chiusi, si possono chiudere anche con spirito umanitario. Potrei dire molte altre cose, ma temo che il tempo sia trascorso. Sui controlli, l'Europa come vuole spendere i 35 miliardi che ha stanziato? I 21 miliardi alle frontiere sono per chiuderle

Abbiamo dunque proposte: vogliamo sollecitare Avramopoulos a dire che il problema è europeo e non italiano e c'è il coro che abbiamo sentito, con il capogruppo del PPE Weber che ha dichiarato che si tratta di un problema europeo e non italiano. C'è molto da fare e l'emergenza c'è, perché spendere 5 miliardi in Italia per avere i risultati di San Ferdinando e Foggia vuol dire che c'è un'emergenza con soldi sprecati e con affarismi dilaganti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Concludo, Presidente, dicendo che non c'è nulla di umanitario nell'aiutare trafficanti che lucrano sulla disperazione dell'Africa; non c'è nulla di umanitario nell'auspicare ed applaudire sbarchi che poi preparano lo schiavismo delle campagne pugliesi o calabresi, perché poi quello succede dopo gli sbarchi. È umanitaria la solidarietà possibile che l'Italia ha sempre praticato, ma con la sicurezza necessaria, che per noi è indispensabile.

La situazione è critica e, a nostro avviso, lei ha agito nel migliore dei modi. Mi scuso in anticipo se userò la seconda persona plurale nel rivolgermi a voi o la prima persona plurale per indicare noi, ma sappia che avrà sempre il nostro appoggio, fino a quando continuerà ad agire in questo modo, mettendo *in primis* il rispetto e la tutela della vita umana, perché così avete fatto; e se così continuerete a fare, avrete il nostro appoggio. La situazione è critica, ma è stata gestita bene: c'era una nave che non si trovava in acque internazionali di competenza italiana e c'erano delle autorità che sarebbero dovute intervenire, ma non lo hanno fatto. Abbiamo fatto il possibile per garantire la sicurezza di queste persone, attraverso la Marina militare e le altre autorità, e non è successo nulla di cui ci si possa incolpare, quindi su questo siamo assolutamente tranquilli. Siamo riusciti però a fare una cosa grandiosa, cioè a sollevare la questione

È importante, questo: siamo riusciti a sollevare la questione politica a livello internazionale ed è giusto che lo si continui a fare. Siamo stati accusati da diversi Paesi di aver agito in modo cinico e crudele - sono stati addirittura usati termini che non voglio ripetere in quest'Aula stesse autorità che in passato hanno agito invece contro la vita umana, con i respingimenti a Ventimiglia, Bardonecchia e in altri luoghi. Dobbiamo far sì che queste cose vengano quantomeno riconosciute,

Ringraziamo i cittadini, le persone, le associazioni e le fondazioni che aiutano in prima persona questi popoli che arrivano in Italia e hanno bisogno di un primo soccorso. Ringraziamo tutti,

grazie.

Ebbene, dobbiamo farlo tutti insieme: andiamo a parlare con tutti i Paesi europei per capire quali sono queste azioni. La diplomazia sicuramente sarà un lavoro estenuante, ma sappiamo di essere in grado di farlo e lo faremo. Vorrei ricordare

Presidente, non mi dilungo troppo, ma facciamo il possibile affinché l'Unione europea venga preservata e si agisca in modo sempre coerente, leale e preciso, facendo in modo che nessuna vita umana sia messa in pericolo. Continuiamo su questa strada, grazie.

Gentile Presidente, onorevoli colleghi, i recenti fatti di cronaca avvenuti in Trecastagni, Comune della provincia di Catania, hanno suscitato allarme e preoccupazione all'interno della cittadinanza, e non solo. Mi riferisco in particolare alle vicende che hanno portato allo scioglimento per mafia del Consiglio e della Giunta del Consiglio e della Giunta comunale, lo scorso 8 maggio, conseguenza inevitabile di quanto emerso dalle attività investigative svolte, alla fine dello scorso anno, dai commissari della prefettura, nell'ambito della cosiddetta inchiesta Gorgoni. L'attività investigativa, durata tre mesi, ha accertato il comportamento infedele di un dirigente e di un funzionario del Comune, i quali, nell'ambito delle procedure volte all'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, avrebbero in più occasioni favorito un imprenditore ritenuto dagli inquirenti vicino ad ambienti malavitosi. Risulta, tra l'altro, che uno dei soggetti interessati sia ritornato in servizio, anche se destinato ad altro ufficio. A tale gravissima circostanza hanno fatto seguito ulteriori avvenimenti, che hanno contribuito ad accrescere la preoccupazione della cittadinanza Presidente, mi potrei fermare qua. Credo che sia poco educativo questo atteggiamento, che si ha puntualmente, quando un senatore - un collega - parla o svolge una relazione di qualsiasi tipo. Sono un'insegnante: ospitiamo spesso delle scolaresche, a

Mi permetto di dire che si educa con la vita e non con le parole: vado avanti. Come dicevo, a tale gravissima circostanza hanno fatto seguito ulteriori avvenimenti, che hanno contribuito ad accrescere la preoccupazione della cittadinanza. In particolare, lo scorso 18 maggio - è questo l'avvenimento particolare a cui vorrei dare risalto, che la stampa,

lasciando evidenti tracce della natura dolosa del gesto compiuto, quasi a voler lanciare un chiaro messaggio al destinatario della loro azione criminale. Si è trattato di un atto di intimidazione contro la Chiesa, in un Sud dove sono assenti le istituzioni, dove il folklore religioso si sposa spesso con la mentalità mafiosa, e dove si minimizza il valore del bene pubblico.

che concorrerebbe a dare un chiaro segnale di vicinanza dello Stato. Non meno incisivo potrebbe essere un intervento di restauro della chiesa, che concorrerebbe a dare agli abitanti un segnale di speranza, in virtù di soluzioni volte a ristabilire lo splendore di Trecastagni, Comune alle pendici dell'Etna.

presto la voce dell'amministrazione comunale, la voce della sindaca, perché è Roma il nostro interesse principale, in questo momento. La preoccupazione è per la nostra città, la nostra capitale e il rischio gravissimo è quello di un nuovo blocco della ripresa economica, che è certamente legata alla rinascita dell'edilizia e agli investimenti privati. Il nuovo stadio è una delle grandi opere che potrebbero contribuire alla ripresa dell'occupazione in questa città. Sotto il Campidoglio pochi giorni fa c'è stata una grande manifestazione dei sindacati che chiedevano lo sblocco delle opere in questa città, quindi la nostra preoccupazione è anche quella di riuscire a ricostruire, a dare una risposta alla grande disoccupazione presente a Roma, che purtroppo è stata travolta dal blocco dell'edilizia.

Ascoltiamo sicuramente con attenzione tutte le voci che verranno su questo, ma ricordiamoci che la ripresa della Capitale deve essere per tutti una priorità